L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: «Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato». Per tale votazione, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un nome. Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età. Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori immediatamente prima dell'ingresso in cabina riceveranno la scheda che dopo il voto depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa. La chiama sarà svolta in rigoroso ordine alfabetico ad eccezione di alcuni pochi colleghi che hanno chiesto di votare per primi. Dichiaro

Complimenti: cresce - ed è di buon auspicio in questi giorni - la presenza femminile nella Presidenza del Senato, con tre Vice Presidenti su

alle quali risponderà il Presidente del Consiglio dei ministri. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

e a quelle che a causa di abusi soffrono in silenzio e non vedono un futuro. *(L'Assemblea si leva in piedi). (Applausi).* Presidente Meloni, lei è la prima Presidente del Consiglio donna nella storia della nostra Repubblica. Sono certo - ce lo ha dimostrato concretamente - della sua straordinaria sensibilità su questo tema. Il valore delle donne è qualcosa di unico, rispettarle non è solo un dovere, ma un imperativo morale. Siamo noi uomini i primi a dovercene rendere conto. Tocca a noi, a tutti noi, fare rumore per tutelare la dignità e il valore delle donne, che passa anche attraverso due binari: il lavoro e la maternità. Gli impegni assunti in campagna elettorale dalla nostra coalizione di centrodestra in materia di lavoro stanno trovando ampiamente riscontro nelle azioni compiute dall'attuale Governo. Da quando lei, presidente Meloni, si è insediata, sono oltre mezzo milione i i posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili. Le cifre positive ci confermano che siamo sulla strada giusta. Siamo però altrettanto consapevoli che non possiamo e non dobbiamo fermarci qui. Le donne, infatti, spesso devono scegliere tra il realizzarsi in ambito professionale - ambizione assolutamente legittima, perché è la premessa per affermarsi anche nella nostra società - e il desiderio di famiglia e di mettere al mondo dei figli, diventando mamme. Dare la vita è qualcosa di unico, di straordinario. D'altronde, come diceva il poeta francese Christian Bobin, gli uomini reggono il mondo, le madri, le donne reggono l'eterno, che regge il mondo e gli uomini. Investire sulla natalità e sulla maternità vuol dire investire sulla vita e sul nostro futuro. Come ha giustamente evidenziato lei, Presidente, agli stati generali sulla famiglia, le donne non sono libere, se devono scegliere tra lavoro, ambizioni professionali e famiglia. Per questo motivo oggi in Senato ho inteso accendere i riflettori su una questione che mi sta molto a cuore: la tutela delle donne passa certamente attraverso le misure di contrasto alla violenza di genere

abbiano consentito in questi tredici mesi l'aumento dei posti di lavoro e del tasso di occupazione. Chiediamo, inoltre, di sapere quali siano le iniziative finora intraprese per invertire l'andamento sulla natalità e quali possano essere i prossimi passi previsti nel proseguo della legislatura.

sede di approvazione delle norme di contrasto alla violenza contro le donne. *(Applausi)*. Ciò dimostra, al di là delle pur numerose polemiche che sempre ci accompagnano, che esiste un terreno sul quale siamo in grado di lavorare insieme e vorrei dire che su questo terreno in particolar modo saremo sempre

che il mercato del lavoro italiano evidenzia rispetto alla media europea hanno rappresentato fin dall'inizio del nostro lavoro una priorità per il Governo, che è intervenuto da subito con misure di stimolo dell'occupazione. E i risultati che abbiamo conseguito stanno di fatto dando ragione a quella impostazione. Le politiche portate avanti in Italia dal 2012 in poi avevano di fatto prodotto un consolidamento del *gap* con le principali economie europee: penso alla dinamica salariale, con gli stipendi che in Italia tra il 2012 e il 2022 diminuivano

che faceva registrare *trend* di crescita molto lenti rispetto al resto d'Europa. Curiosamente, nello stesso periodo si registrava anche una mobilitazione abbastanza contenuta anche...

Dicevo che si registravano *trend* di crescita molto lenti rispetto al resto d'Europa. Ma con l'attuale Governo è cambiata l'impostazione che guida gli interventi in tema di lavoro, che ora sono volti soprattutto a incentivare l'occupazione e a garantire più soldi in busta paga, soprattutto attraverso il taglio del cuneo contributivo. Penso all'attenzione che anche in questa manovra economica abbiamo messo sul tema dei rinnovi contrattuali. Devo dire che questo ha portato anche un cambio di atteggiamento da parte di alcune organizzazioni sindacali, che prima avevano una mobilitazione abbastanza contenuta: ho registrato tra il 2012 e il 2022 circa sei scioperi generali, mediamente uno ogni due anni, mentre adesso se ne fanno due ogni anno e anche questa è una buona notizia.

*record* del tasso di occupazione, *record* di occupati e occupati permanenti, oltre mezzo milione di lavoratori in più, di cui 443.000 stabili, *record* di occupazione femminile in termini assoluti e di tasso di occupazione. Per quanto attiene in particolare al tema del lavoro femminile, credo che questi risultati siano anche il frutto di misure che hanno hanno avuto l'obiettivo di incentivare l'occupazione, soprattutto favorendo tempi di vita e tempi di lavoro, cioè non costringere le donne - come l'interrogante diceva correttamente - a dover scegliere, perché quello non vuol dire avere libertà. Si ha la libertà se si ha la libertà di fare tutte

favorire il lavoro delle mamme. E sono interventi che seguono quelli già realizzati, li potenzieremo, ne affiancheremo di nuovi, speriamo anche con il contributo del Parlamento. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare affinché il mercato del lavoro italiano continui questa sua tendenza positiva che però - senatore De Poli - per i dati e, particolarmente per i dati che riguardano il lavoro femminile, è forse il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di Governo.

È un fatto veramente importante il riferimento soprattutto al potenziamento rispetto a quello che sarà il prossimo futuro, con un'attenzione verso l'occupazione nel suo contesto generale e, in modo particolare, per quello femminile. *(Applausi)*.

Cb))*. Signora Presidente del Consiglio, in diverse occasioni le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno richiamato l'attenzione del Governo sull'erosione delle loro competenze a seguito della riforma costituzionale del 2001. Ad essere tradito è stato lo spirito stesso della riforma. Per le autonomie speciali avrebbe dovuto portare

Si è sedimentato invece un orientamento centralista, confermato dal susseguirsi di impugnazione delle leggi regionali e provinciali e dalle sentenze della Corte costituzionale. Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano il ripristino delle competenze è anche una questione di diritto internazionale. Fu il livello di autonomia raggiunto nel 1992 a convincere l'Austria a rilasciare la quietanza liberatoria, mettendo fine alla controversia internazionale sollevata nel 1960 all'ONU. È un tema sul quale lei si è espressa anche nel suo discorso di insediamento, annunciando un preciso impegno per il ripristino degli *standard* di autonomia del 1992. Anche per questo lo scorso ottobre il presidente Kompatscher, in qualità di coordinatore delle autonomie speciali, le ha consegnato una proposta di legge costituzionale, che mira a definire i limiti alle rispettive competenze di Stato, Regioni e Province speciali e a introdurre il principio dell'intesa per le modifiche future degli Statuti di autonomia. Come specificato nella relazione illustrativa, si tratterebbe non di un completo adeguamento degli Statuti, ma di un primo passo in attesa di una riforma generale del sistema delle autonomie speciali. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se lei non intenda sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri il testo proposto dai Presidenti delle autonomie speciali, affinché sia fatto proprio in un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa. In tal caso si chiede quali tempistiche è in grado di prevedere per l'avvio formale dell'*iter* di approvazione dello stesso in modo che possa essere successivamente avviato l'*iter* approvativo anche da parte dei Consigli regionali interessati. La ringrazio, signor Presidente. (Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna) e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale i proponenti chiedono di modificare i rispettivi Statuti speciali in un quadro condiviso con lo Stato. In coerenza con l'attenzione che questo Governo attribuisce al tema dell'autonomia regionale, a quello delle valutazioni sul ripristino delle competenze modificate dalla riforma del 2001, i contenuti del testo trasmesso sono ora in corso di approfondimento tecnico e sono in ogni caso oggetto di particolare attenzione da parte nostra. Le preannuncio in proposito che è mia intenzione promuovere l'avvio di tavoli di confronto bilaterale con ciascuna delle quattro Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per poter insieme valutare tutte le necessarie iniziative da parte del Governo. Si richiama il principio per cui, ad oggi, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla riforma costituzionale del Titolo V, trova applicazione la clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sulla base dell'interpretazione che in questi anni ne ha dato la Corte costituzionale. Con riferimento alla procedura di revisione degli Statuti, l'iniziativa dei Presidenti di Regione e delle Province autonome citate intende introdurre, in luogo del parere del Consiglio regionale e provinciale, il principio il principio dell'intesa, prevedendo che sul testo delle leggi costituzionali di revisione degli Statuti, approvato in prima deliberazione dalle Camere, sia acquisita l'intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e provinciale, prevedendo la decadenza della proposta di revisione nel caso di mancato raggiungimento della medesima intesa nel termine di tre mesi. Sul punto il Governo intende approfondire questa ipotesi in spirito collaborativo. Siamo aperti e voglio dirle di più: abbiamo il vantaggio di poter contare, con riferimento alle interlocuzioni sopra richiamate, sulla specifica sensibilità e sulla specifica attenzione maturata dal ministro per gli affari regionali e le autonomie di questo Governo, Roberto Calderoli, che nella scorsa legislatura - come lei sa - è stato Presidente della Commissione paritetica per Bolzano e componente della Commissione paritetica per il Trentino-Alto Adige. Quindi mi pare che siamo in ottime mani.

nel 1992; anche per questo ci siamo astenuti e non abbiamo votato contro il suo Governo. Devo dire che la sua risposta è soddisfacente in parte, perché tutti sappiamo che l'*iter* di una legge costituzionale è molto complesso e impegna molto tempo; pertanto penso che tutta questa procedura dovrebbe essere accelerata, per arrivare ancora in tempo e

finestra") sulla crescita economica del Paese e le politiche congiunturali, chi avesse sentito, in Aula o tramite la televisione, la sua risposta al collega De Poli avrebbe l'impressione che viviamo in un Paese straordinariamente in crescita. Mi provo a mettere nei panni del cittadino che l'ascolta da casa. Lei è qui al Governo da più di un anno. Nell'ottobre del 2022 la benzina costava 1,6 euro al litro e oggi costa 1,9 euro. I trasporti sono aumentati del 7

non corrisponde alla realtà del Paese. Lei, signora Presidente, ha vinto le elezioni con il 26 per cento, grazie a una straordinaria prova di coerenza della quale dobbiamo darle atto. Lei era all'opposizione, mentre noi avevamo da sostenere il peso del Governo Draghi e prima ancora del Governo della pandemia. Lei giustamente, dal suo osservatorio, lucrava il consenso sbandierando la bandiera della coerenza. Oggi non c'è un solo argomento sul quale ella stia dimostrando coerenza. Aveva detto che avrebbe bloccato l'immigrazione e che avrebbe chiuso i porti: gli sbarchi sono raddoppiati e l'unico blocco è quello del rientro della fuga dei cervelli. Aveva detto alla Germania (me lo ricordo, perché facevo un altro lavoro e anche lei ne faceva un altro) che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo dovuti uscire dall'euro. Ieri l'ho vista in tutt'altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso *spot*, del quale voglio darle atto (straordinaria attrice), che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei ha aumentato, rispetto al Governo Draghi, le accise sulle benzina. Potrei continuare sulle trivelle e su tante altre questioni. Il punto politico è che la sua coerenza, signora Presidente, si è fermata al momento in cui è stata all'opposizione. Non le parlo, per carità di patria, di giustizia, che purtroppo - lo dico al mio Ministro preferito ormai in tv è a "Chi l'ha visto", perché la riforma della giustizia non la vede più nessuno. Non le parlo, per carità di patria, nemmeno del tema del PNNR, in larga parte basato sul ruolo delle ferrovie, dei trasporti e delle infrastrutture, ma oggi non mi sento di maramaldeggiare. Le chiedo, signora Presidente, se può indicarci tre punti su cui, da qui al 2024, è in grado di cambiare la logica economica di questo Paese, atteso che ha raccontato che va tutto bene, ma il ceto medio, da quando c'è lei - sarà sfortuna, sarà casualità - paga molto caro il prezzo

la situazione di questa Nazione rispetto alla condizione nella quale l'abbiamo trovata. Con tutto il rispetto, guardi che non lo dico io: penso che sia sotto gli occhi di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia, per esempio, degli investitori e dei mercati nell'economia italiana.

comprino molto volentieri i nostri titoli di Stato, che lo *spread* sia ai minimi da molto tempo *(Applausi)* e che la Borsa italiana cresca più di quanto crescano tutte le altre borse europee europee siano dati che dicono qualcosa di più rispetto alle valutazioni - legittime, ovviamente - dell'opposizione. E guardi che lo abbiamo fatto in piena coerenza,

Poi non abbiamo la bacchetta magica per fare i miracoli, perché, per esempio, il costo della benzina, come sa, dipende soprattutto dalle scelte che fanno i Paesi che detengono il petrolio: se ci volesse dare una mano con il suo amico Mohammad bin Salman *(Applausi)*, forse ci aiuterebbe ad abbassare il prezzo della benzina.

anni e anni che l'Italia non cresceva più della media europea. Penso che anche questo sia importante. Francamente, mi ha lasciato un po' stupita che nell'interrogazione abbiate il rimbalzo del PIL nel biennio post-Covid come se fosse un parametro di riferimento. Senatore Renzi, lei, che è una persona seria e capace, saprà è cresciuta più di altri nel 2021 e nel 2022 banalmente perché la sua economia era tracollata durante il Covid *(Applausi)*, nonostante i 180 miliardi di euro spesi

L'Italia è stata tra i primi in Europa a ottenere fondi. Le uniche difficoltà che abbiamo riscontrato sono relative a obiettivi che avevamo ereditato (penso allo stadio di Firenze: ho ascoltato anche le sue critiche, per la verità un po' tardive), ma quello che abbiamo fatto è stato cercare di fare in modo che le risorse non andassero disperse per progetti che non erano finanziabili, né realizzabili *(Applausi)*, perché vogliamo mettere a terra quelle risorse. Penso che si vedrà anche nelle prossime ore il lavoro molto proficuo che stiamo facendo con la Commissione europea, ma, anche in questo caso, l'auspicio di certa opposizione che ha tifato contro l'Italia sperando che le rate non venissero pagate purtroppo finora è stato tradito. vederla cambiare in questo modo. Lei ci raccontava dall'opposizione di quanto la voce del popolo dovesse essere ascoltata. Io le ho parlato di riso, zucchine, pane e pasta e lei si è messa a parlare dello *spread*, si è messa a parlare di quanto è lo *spread*, dicendo che è più basso di prima. Stia tranquilla, stia serena: è molto più basso di quello che avevamo noi, ma non è questo il punto. Signora Presidente, noi siamo qui per aiutarla rispetto alle sue evidenti difficoltà. Vede, signora Presidente, ci siamo passati tutti: quella seggiola lì, quella accanto, si è abituati ad avere intorno un coro di adulatori che ti dicono bravo, i *laudatores* che ti fanno gli applausi e uno tende a crederci alle cose che dice. Lei viene in Parlamento e qualcuno le chiede una indicazione per darle una mano, persino sul petrolio. Io per il mio Paese le do una mano su qualsiasi cosa e lei lo sa. Ci sono centinaia di SMS a dimostrarlo. Il punto non è quello, cara Presidente del Consiglio. Il punto è che lei si trova a guidare un Paese non con lo stile di una che fa la campagna all'opposizione, ma con il fatto che non sta governando la situazione economica delle famiglie. Allora le dico, con molta tranquillità, che, lei ha voglia di venire in Parlamento e pensare di raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e continua a fare tutto bene, vada avanti, avrà un risveglio - se lo faccia dire da un esperto della materia - terribile. Il punto centrale è che lei in questo momento, cara Presidente del Consiglio, si trova a che fare con un racconto di sé stessa secondo il quale lei sarebbe la povera Cenerentola. Ma lei non è né Cenerentola, né la bella addormentata nel bosco, né Biancaneve e i sette nani. È la Presidente del Consiglio dei ministri che non ha fiducia nella sua squadra e che vede, mai come in questo momento, aumentare la benzina, il costo della vita e la qualità delle persone.

politiche di tutela contro gli eventi climatici estremi e per la messa in sicurezza del territorio, dell'osservatorio CittàClima, nel 2022 nel nostro Paese sono aumentati del 55 per cento gli eventi meteo idrogeologici rispetto al 2021, con 310 fenomeni meteorologici che hanno provocato danni ingentissimi e addirittura 29 morti. È un'emergenza che quest'anno - come tutti sappiamo - ha riguardato innanzitutto l'Emilia Romagna, duramente colpita dall'alluvione del maggio scorso, che ha provocato 16 morti e una perdita economica stimata in quasi 9 miliardi di euro. È stata la terza catastrofe naturale più dannosa al mondo nel primo semestre dell'anno. In quel caso furono duramente colpiti 44 Comuni romagnoli e, secondo una stima parziale, la metà dei danni riguarda fiumi, strade e infrastrutture pubbliche per oltre quattro miliardi di euro e privati per oltre 1,2. Il 21 maggio, Presidente, lei ha promesso che il Governo avrebbe dato massima priorità all'uscita dall'emergenza, alla completa ricostruzione e al tempestivo ritorno alla normalità delle zone colpite. colpite. Dopo sei mesi, però, nonostante quei proclami, le famiglie sfollate che hanno perso tutto hanno ottenuto soltanto un acconto di 3.000 euro e tutti - privati e aziende - sono ancora in attesa delle risorse che erano state promesse. Solo qualche giorno fa, con un ritardo davvero colpevole e clamoroso, il 15 di novembre, è stata attivata la piattaforma informatica cui inviare le richieste di ristoro. Naturalmente quella dell'Emilia Romagna non è stata purtroppo l'unica alluvione: tra il 15 e il 16 settembre furono colpite le Marche. In quel caso ci furono 13 vittime e 50 feriti. Situazione analoga è quella abbattutasi in Campania nell'isola d'Ischia, Comune di Casamicciola, la mattina del 26 novembre del 2022. Anche in quel caso ci furono 12 vittime, 5 feriti e persone sfollate. Invece è ancora troppo presto per quantificare i danni derivanti dall'alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso novembre, ma anche in questo caso parliamo di danni molto seri. Signora Presidente, siccome questi eventi sono sempre più frequenti, peraltro su un territorio come quello italiano, caratterizzato da una elevatissima esposizione al rischio idrogeologico e anche a quello sismico, io le chiedo i motivi di tutto questo ritardo nei ristori destinati ai territori citati. Soprattutto, signora Presidente, le chiedo quali attività concrete intende compiere il Governo per provare, finalmente, a mettere in sicurezza il territorio,

De Cristofaro, per quello che riguarda l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, la ringrazio per darmi l'occasione di questa risposta, perché il Governo - come si sa - ha assunto, all'indomani dell'alluvione, misure eccezionali, immediate, che vale la pena di ricordare. Con il decreto n. 61 abbiamo prima stanziato quasi 1,8 miliardi per la tenuta del sistema produttivo e i livelli occupazionali; con il decreto n. 88 abbiamo stanziato altri 2,5 miliardi per la ricostruzione pubblica, oltre 120 milioni per i primi contributi alla ricostruzione privata e 100 milioni per le imprese. A queste risorse si sono aggiunti altri 149 milioni con successivo provvedimento. Con il lavoro del commissario Figliuolo, dei 2,5 miliardi stanziati per la ricostruzione pubblica con il decreto n. 88, è già stata messa a disposizione degli enti locali una somma pari a 1,445 miliardi, tra interventi per somme urgenze, messa in sicurezza idraulica e infrastrutturazione varie. A queste risorse se ne aggiungono altre, non inferiori al miliardo, già nella disponibilità del Commissario. Sono stati poi già erogati 100 milioni alle famiglie per il sostegno immediato e il contributo di auto sistemazione; 60.000 giornate di cassa integrazione; 200 milioni per i lavoratori autonomi; altri 600 milioni sono già nella disponibilità del Commissario. Ai 4,5 miliardi di euro stanziati con i decreti nn. 61 e 88, si aggiungeranno altri 700 milioni di credito d'imposta previsti dalla manovra e poi le risorse messe a disposizione dei vari Ministeri, tra cui gli oltre 150 milioni di euro del Masaf per ripagare i danni del settore agricolo. Approfitto dell'occasione anche per annunciare che, nell'ambito della revisione del PNRR, della quale parlavamo poc'anzi, il Governo ha proposto un intervento per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, colpite dall'alluvione nel maggio scorso, pari a un ulteriore 1,2 miliardi di euro; risorse di euro; risorse che consentiranno anche di utilizzare le deroghe e le semplificazioni del PNRR. Se non vado errata, facendo un conto a spanne, siamo a 6,5 miliardi Quindi, non ci sono nessuna promessa mancata e nessuna distrazione, almeno non da parte del Governo, perché, anche qui - mi consenta di segnalare, sommessamente - che la piattaforma Sfinge, di competenza della Regione Emilia-Romagna, cioè lo strumento attraverso il quale i privati possono presentare le domande di risarcimento, è operativa solo dal 15 novembre scorso: due mesi dopo l'ordinanza del Commissario, che è del 14 settembre. che, senza la piena operatività della piattaforma, è impossibile trarre la quantificazione precisa dei danni e la definizione dell'ulteriore fabbisogno finanziario, compreso per quanto riguarda i beni mobili. Aggiungo che il Governo sta ancora aspettando dalla Regione anche il quadro complessivo delle criticità esistenti prima delle alluvioni e delle opere che sono state realizzate per metterlo in sicurezza. È una ricognizione necessaria, anche questa, per rassicurare i cittadini. Per cui, come vede, il Governo ha agito con il massimo sforzo, senza polemiche, guardando ai bisogni dei cittadini e non al colore politico dell'interlocutore istituzionale. Devo dire, però, che mi rendo conto che questo non è un costume particolarmente diffuso. Dopodiché, noi continuiamo a lavorare anche in tema di messa in sicurezza del territorio, dove lei sa che vi sono soprattutto risorse del PNRR, disponibili e salvaguardate. Questo sarà oggetto - ovviamente è già oggetto - del lavoro che sta svolgendo particolarmente il ministro Musumeci e che porteremo avanti nei prossimi mesi. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica

oppure c'è una mancata volontà di comprendere e di ostinarsi a non capire che in questo Paese sono totalmente cambiate le priorità?

ha detto tante volte in queste settimane che nel suo Governo non ci sono negazionisti climatici. Eppure, siete lenti nei ristori e vi rifiutate di discutere della necessità di una legge sul clima e di una legge sul suolo. Vi ho chiesto anche cosa intendete fare per il futuro,

che in Europa hanno votato contro la legge per il ripristino della natura. Conducete una lotta senza quartiere all'auto elettrica e all'efficientamento energetico delle case. Tutto ciò senza comprendere che questa ideologia, davvero antistorica, ridurrà a brandelli la capacità industriale dell'Italia. E fate lo stesso nella manovra finanziaria e ve lo diremo nei prossimi giorni. Signora Presidente del Consiglio, almeno non offendetevi se qualcuno, come facciamo noi

*(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente del Consiglio, fin dal giorno del suo insediamento il suo Governo ha avviato un percorso riformatore e lo ha fatto con serietà, con senso di responsabilità e visione. Ha parlato chiaro, spiegando ai cittadini quali fossero le difficoltà, quali le opportunità e lo ha fatto in modo che le difficoltà non soffocassero le fasce più deboli di un'Italia piegata dopo la crisi post pandemica ed energetica. Già dalla legge di bilancio dello scorso anno, come in quella che ci accingiamo ad approvare a dicembre, abbiamo impegnato le risorse in due direzioni ben precise. La prima è, da un lato, la tutela delle famiglie con i redditi più bassi attraverso il *bonus* sociale elettrico e gas; dall'altro, si fronteggia l'aumento dell'inflazione con la *social card* "Dedicata a te". Tutto questo guardando e preoccupandoci degli ultimi, contrastando la povertà, tutelando chi ha lavorato una vita intera e merita una pensione dignitosa, e tutelando chi davvero non può lavorare attraverso l'assegno di inclusione. Per chi invece può farlo, abbiamo avuto il coraggio di superare l'assistenzialismo a fini elettorali e di avviare un sistema di attivazione del lavoro e della formazione. La seconda direzione verso la quale abbiamo indirizzato la nostra azione è la messa a terra di quelle riforme in grado di rilanciare la crescita. È in quest'ottica che abbiamo ridotto e confermato per il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale fino al 7 per cento, garantendo così più soldi in busta paga per 14 milioni di lavoratori e importanti vantaggi per le imprese che assumono, in modo da creare un circolo virtuoso che farà da stimolo per l'economia. delle partite IVA, innalzando da 60.000 a 85.000 euro il limite per entrare nella *flat tax* al 15 per cento. La riforma di cui tutti abbiamo bisogno è quella fiscale, fondamentale anche per combattere l'evasione. Con la riduzione da quattro a tre delle aliquote Irpef, il Governo ha compiuto il primo passo per avviare il grande e ambizioso progetto di pagare meno, ma pagare tutti. Con il concordato preventivo e la delega fiscale si dà vita a un nuovo e più costruttivo rapporto tra fisco e contribuenti. Né possiamo ignorare i grandi investimenti di questo Governo sulla sanità la particolare attenzione - lo diceva prima - alle politiche per la natalità, attraverso l'aumento dell'assegno unico per i figli, e per il congedo parentale, che passa dal 30 all'80 Fin qui, signor Presidente, è il grande lavoro fatto in poco più di un anno. Quindi, diversamente dalla logica distruttiva che abbiamo ascoltato fino ad ora, le chiediamo quali saranno i prossimi passi che il Governo vorrà fare per famiglie e lavoratori, e per proseguire la strada verso la riduzione della pressione fiscale.

per famiglie e imprese siano stati dall'inizio una priorità di questo Governo. È una visione che avevamo già intrapreso con la legge di bilancio 2023, che confermiamo con la manovra di bilancio 2024 e che provo a sintetizzare anche io.

di reddito in un unico scaglione al quale si applica l'aliquota del 23 per cento, con un risparmio annuo che arriva fino a 260 euro; l'aumento della soglia di detassazione dei *fringe benefit* dagli attuali 258 euro fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro per tutti gli altri; il dimezzamento della tassazione sui premi di produttività; la diminuzione del canone in bolletta da 90 a 70 euro. Abbiamo poi introdotto un pacchetto di misure dedicate alle famiglie con figli: come sapete, si prevede l'esonero completo dal pagamento dei contributi per le lavoratrici dipendenti stabili con due figli fino al compimento dei dieci anni del figlio più piccolo e con almeno tre figli, fino al compimento dei del figlio più piccolo. Credo sia un segnale estremamente importante. L'esonero ha un limite massimo annuo di 3.000 euro e corrisponde anche al beneficio lordo annuo in busta paga. l'aumento del *bonus* nido a 3.600 euro annui per i nati nel 2024 con almeno un fratello *under* dieci per famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. La mensilità aggiuntiva di congedo parentale retribuita al 60 per cento per quest'anno è all'80 Per le imprese, abbiamo introdotto una superdeduzione del 120 per cento del costo del lavoro in caso di nuove assunzioni, purché si tratti di maggiore occupazione, quello che chiamiamo il "più assumi meno paghi", che arriva al 130 per cento se si assumono mamme, giovani, disabili, ex percettori di reddito di cittadinanza. Per i lavoratori autonomi, dopo l'estensione del regime forfettario, abbiamo rinviato al 2024 l'acconto Irpef di novembre, consentito la rateizzazione anche fino a cinque mesi e abbiamo introdotto il concordato preventivo preventivo biennale. È un lavoro che chiaramente racconta una visione, che va fatto immaginando una legislatura che è quella che abbiamo a disposizione per cercare di fare sempre dei passi avanti. Il prossimo passo da compiere la completa attuazione della delega fiscale, che chiaramente scandirà gli ulteriori prossimi passi in questo senso e dopo un'attesa durata decenni consentirà finalmente di riformare profondamente il fisco italiano, rendendolo più giusto, più efficiente e capace di fare la sua parte nel ricostruire il rapporto che serve tra lo Stato e gli italiani, che noi non consideriamo sudditi, ma vogliamo considerare cittadini. *(Applausi)*.

prestabilita fin dall'inizio. Sapevamo che non sarebbe stato facile, sapevamo che oltre alle difficoltà da affrontare per rimettere in ordine i conti e arginare la crisi, avremmo avuto a che fare anche con una falsa narrazione. Per questo abbiamo smontato questa propaganda e la *fake news* in base alla quale avremmo aumentato la pressione fiscale: bastava leggere la manovra di bilancio per rendersi conto che questo Governo le tasse non le ha alzate, anzi le abbassa per quei 14 milioni di italiani che potranno puntare su 100 euro in più in busta paga. *(Applausi)*. Le abbassa e continuerà a farlo, fatevene una ragione. Questo a differenza di qualcun altro che l'ha preceduta, signor Presidente, che invece di raccontare la verità ai cittadini ha fatto leggi di bilancio lacrime e sangue, favorito la disoccupazione con il reddito di cittadinanza, dissanguando i conti del Paese. *(Applausi)*. Soltanto il nostro senso di responsabilità e la competenza di questo Governo riusciranno a risanarli, senza far pagare le spese agli italiani. C'è una cosa che per il centrodestra è sacra ed è l'impegno

rispetto al conflitto in Ucraina e alle principali crisi inte[...]

chi lei riteneva fosse il Presidente dell'Unione africana. Non mi soffermo sul quel contesto, perché è stato detto tutto in queste settimane, come pure non credo sia questo il contesto in cui chiedere come sia potuto accadere, anche se ovviamente è una domanda che ci interessa; rischieremmo però di rendere labile il confine tra elementi di grande preoccupazione per l'interesse e la sicurezza nazionale ed elementi tragicomici, modello ambasciatore del Catonga. Preferisco invece entrare nel merito delle cose che lei ha detto in quella telefonata, perché, devo dire la verità, la Meloni al telefono ci è piaciuta molto, ha detto delle cose che riteniamo giuste e importanti, quelle che stiamo dicendo noi del MoVimento 5 Stelle da molti mesi. Lei ha detto bisogna trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti e noi riteniamo che sia davvero la strada da percorrere. Però c'è una Meloni al telefono e una Meloni in presenza, quella che invece nelle Aule parlamentari e in consessi internazionali dice il contrario. A dicembre ironizzava sul fatto che noi dovevamo proporre il reddito di cittadinanza ai russi per farli ritirare, ma il 13 maggio disse di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina; rispetto alle ricostruzioni di ciò che è accaduto nel vertice G20 di ieri, quando il Putin, il dittatore Putin, dice che dobbiamo mettere fine alla guerra, lei dice che l'unico modo è che la Russia si ritiri. Anche i miei figli si rendono conto che c'è una discrasia enorme tra il sostenere che una via d'uscita accettabile per ambo le parti sia l'unica strada e ritenere, invece, che la Russia deve ritirarsi e che questo sarà l'unico modo per far finire la guerra. La domanda che sorge spontanea è, dunque, qual è la Meloni vera, quella al telefono o quella in presenza? Lei pensa le cose che ha detto quel giorno al telefono o conferma invece la linea che ha mantenuto sempre nei consessi istituzionali?

collega Patuanelli, anche io non torno sulle ragioni e sugli errori che hanno purtroppo consentito a due comici russi di spacciarsi per il Presidente dell'Unione africana; sono state ampiamente oggetto di approfondimento. Utilizzo invece il mio tempo per risponderle molto volentieri sui contenuti della telefonata, banalmente perché io sono fiera di aver dimostrato ancora una volta la coerenza delle posizioni mie e del Governo italiano in tema di politica estera e sono fiera di essere lontana anni luce dal modello di chi prima di me si mostrava condiscendente in privato, salvo poi mostrare i denti a favore di telecamera o votava il sostegno militare a Kiev finché si trattava di mantenere il proprio posto al Governo, per poi decidere di sostenere che Kiev non andasse più aiutata quando è passato all'opposizione per guadagnare consenso facile. *(Applausi)*. In questo caso, però, questo consenso facile si guadagna sulla pelle e sulla libertà di una Nazione sovrana. In quella telefonata ho detto quello che tante volte ho ripetuto anche in questo Parlamento. primo, che noi siamo a fianco dell'Ucraina, ribadendolo anche in quella telefonata. Ho detto che cerchiamo una pace giusta in linea con il diritto internazionale e che siamo pronti a fare le nostre proposte, che chiaramente, nel caso, confronteremo anche con il Parlamento quando dovessero esserci i margini per quella pace giusta. Il punto sul quale io, lei e voi non ci capiamo per arrivare a un'opzione di questo tipo, l'unico modo - come io ho detto decine di volte in quest'Aula parlamentare - è mantenere un equilibrio tra le forze in campo, che vuol dire sostenere l'Ucraina *(Applausi)*. Se noi avessimo fatto quello che qualcuno ci chiedeva in questa Aula, e cioè smettere di sostenere l'Ucraina, purtroppo non avremmo avuto una pace, come qualcuno va dicendo in giro: noi avremmo avuto un'invasione e un'invasione non si chiama pace. *(Applausi)*. Io non sono così cinica da scambiare le due due cose. Continuo quindi a ritenere che l'unico modo possibile per arrivare eventualmente anche a una soluzione diplomatica del conflitto è sostenere l'Ucraina. È quello che ho detto in quest'Aula, è quello che faccio, è quello che ho ribadito all'interno di quella telefonata. Questo non vuol dire che io non mi renda conto della difficoltà che è presente anche nella nostra opinione pubblica; ho detto anche questo e anche questo l'ho sostenuto all'interno di queste Aule parlamentari e ciò ha fatto molto discutere. Io sono perfettamente consapevole della stanchezza dell'opinione pubblica perché ascolto la gente, sono capace di farlo. Quello che fa la differenza tra la mia scelta e altre scelte è che io penso che la responsabilità della politica sia guidare la società, non rincorrerla. E non mi stupisce che persone che non hanno gli stessi elementi che ho io per giudicare possano fare valutazioni diverse, che persone che non hanno chiaramente sulla loro spalle le decisioni che che in qualche maniera compromettono il destino di una Nazione possano fare altre valutazioni. Ritengo in coscienza di dover fare le mie per le responsabilità che ho ed è quello che sto facendo. Ma questo non vuol dire che non capisca gli italiani anche quando chiedono se, nella condizione in cui siamo, possiamo davvero permetterci di fare quello che stiamo facendo. Continuerò a essere convinta che noi, aiutando e sostenendo gli ucraini che combattono, stiamo difendendo il nostro interesse nazionale *(Applausi)*. Ho però detto anche in quest'Aula, l'ultima volta che sono venuta prima del Consiglio europeo - se lo ricordate e se siamo intellettualmente onesti che, proprio perché sono consapevole delle difficoltà che le nostre società stanno pagando, noi non potevamo, ad esempio, in Consiglio europeo sostenere la tesi, che pure altre Nazioni sostengono, per la quale la per la quale la revisione del bilancio pluriennale si potesse rivedere solamente per l'Ucraina, e ciò se non eravamo in grado anche di mettere risorse sulle conseguenze che le nostre società stanno pagando per il conflitto in Ucraina. Che cosa ho detto? Ho detto che sono consapevole della situazione per cui, guardi, anche stavolta, a prova di telecamera, non c'è una Meloni in privato e una Meloni in pubblico, quello lo abbiamo visto altre volte. *(Applausi)*. C'è una Meloni che dice sempre quello che pensa, che lo dice con chiarezza e lealtà e che per questo consente all'Italia oggi di essere rispettata e di essere ascoltata come purtroppo non è stata quando la guidavate voi. *(Applausi)*. Signor Presidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è che non ho capito se, quando ci chiedeva di dare 1.000 euro con un *click* a tutti gli italiani, lei stava guidando, subendo o seguendo la società. Non c'è molto tempo per approfondire questo argomento. Devo dire che mi sento parzialmente soddisfatto della sua risposta perché la domanda voleva ovviamente evidenziare le contraddizioni, che sono emerse anche adesso. Lei continua a sostenere che ciò che ha detto in quella telefonata - bisogna trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti - è coerente con il dire che scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Queste due cose sono in totale contraddizione. Ricordo quindi che una volta è stato votato l'invio delle armi. Due settimane dopo lo scoppio della guerra, siamo stati i primi a dire che in quella fase era necessario. Si può avere un'opinione diversa su quale sia la strada. Il problema è che la strada del continuo armamento è un fallimento nei fatti, perché non ha portato alcun risultato. *(Applausi)*. Proviamo un'alternativa. *(Applausi)*. Non siamo certi che smettere di armare l'Ucraina porti automaticamente ma almeno proviamoci. Nel frattempo la gente continua a morire e nel nostro Paese continuano a esserci problemi economici legati a un conflitto molto importante, che è ancora in corso. credo che sia mancata una cosa, e mi dispiace molto, perché in quella telefonata certi elementi c'erano. È mancato il coraggio di dire quelle cose pubblicamente nei tavoli internazionali, perché forse non si vuole infastidire nessun alleato. Credo che si debba invece avere il coraggio di difendere gli interessi della nostra Nazione non nelle telefonate private, ma nei consessi internazionali. E credo che, soprattutto per chi si professa patriota, non farlo sia piuttosto surreale.

che per la Lega il tema della sicurezza è sempre stato centrale nella propria azione politica, fin dai tempi delle esperienze di Governo passate. Ricordo i patti per la sicurezza dell'allora ministro Roberto Maroni, che salutiamo, visto che

non solo azioni repressive, ma anche preventive, di contrasto all'immigrazione clandestina, con risultati a dir poco straordinari. Noi siamo contenti e soddisfatti della politica che il Governo sta portando avanti su questo tema, non solo perché il tema della sicurezza è all'interno del programma elettorale in tutte le sue forme, declinato in maniera molto chiara ed evidente. Ci sono state alcune azioni importanti, come l'adeguamento della dotazione del personale delle Forze dell'ordine. Ci saranno 12.000 persone in più l'anno prossimo: finalmente un impegno che va in questa direzione. Penso inoltre alla norma per cercare di dare una stretta sulle occupazioni abusive all'aggravante di un terzo della pena per chi offende e sostanzialmente aggredisce le Forze dell'ordine, perché la tutela e il rispetto della divisa sono sacrosanti. Parlavamo di rispetto ed è importante anche il rispetto delle istituzioni. Penso alla tutela legale nei confronti delle stesse Forze dell'ordine. Siamo soddisfatti anche perché ci sono alcuni elementi che il Governo ha introdotto che caratterizzano molto l'azione della Lega, e noi di questo le siamo grati. In alcuni decreti - ricordiamo il decreto Cutro - è finita comunque la stretta sulla protezione speciale, un elemento che la Lega ha voluto fortemente, soprattutto nei confronti di quegli immigrati che arrivano da Paesi sicuri e che quindi non si capisce perché abbiano bisogno di una protezione speciale, invece dovrebbero semplicemente essere rimpatriati, se quei Paesi sono considerati sicuri. Ci sono poi le norme legate alla sicurezza urbana; l'istituzione dell'osservatorio sulle periferie, che darà una dimensione reale di tutte le difficoltà che ci sono; il contrasto alla criminalità e alla microcriminalità. del decreto Caivano sono state recepite alcune misure importanti che erano contenute nel nostro disegno di legge per contrastare il fenomeno delle *baby gang*, perché è proprio fra i bulli e i prepotenti che la mafia raccoglie le proprie reclute; quindi contrastare la microcriminalità significa contrastare anche il il grande crimine. Dovremmo ricordarci che questa è un po' la posizione storica del centrodestra, con tutta una serie di misure che sono anche legate all'educazione - mi avvio a concludere - tipo la rieducazione del minore, l'ammonimento del questore, il coinvolgimento delle famiglie (importantissimo), il il rafforzamento dell'obbligo scolastico e, per ultimo, il contrasto alle truffe nei confronti degli anziani. Alla luce di tutto questo chiaramente noi le chiediamo, vista la strada importante che sta aprendo il Governo, quali altri provvedimenti intenda adottare per proseguire con le misure sulla sicurezza,

il Governo ha varato, in questo primo anno, diversi provvedimenti in materia di sicurezza. È un lavoro puntuale che facciamo con convinzione e determinazione. Lo abbiamo fatto e lo facciamo perché garantire sicurezza non ci permette semplicemente - e sarebbe già sufficiente - di difendere i più fragili e soprattutto gli indifesi della nostra società. Alla fine, la sicurezza serve soprattutto a chi è più debole. Ma lo

una grande materia economica. Prendo qui a esempio il dispiegamento di 800 militari nelle stazioni e le norme antiborseggio che abbiamo varato nell'ultimo pacchetto sicurezza, ovvero il divieto di accesso alle metropolitane e alle stazioni per chi è già stato denunciato e condannato per furto, rapina e altri reati contro il patrimonio o la persona che vengono commessi in quei luoghi. Sono chiaramente norme di buon senso, che non servono semplicemente a difendere i cittadini che ogni giorno usano i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro,

i nostri flussi turistici aumentano e questo si traduce in ricchezza e posti di lavoro. Le faccio un altro esempio: le norme contro le occupazioni abusive che abbiamo approvato, come sa, derivano da un'antica battaglia che abbiamo portato avanti. Dire che la proprietà privata è sacra, sacra, che un immobile non si può occupare e che, se lo si occupa illegalmente, la Polizia interviene immediatamente, quando il proprietario ne faccia denuncia, invece di lasciarlo lì ad aspettare per anni, in attesa di vedersi riconosciuto un diritto

la volontà di rendere questa di nuovo una Nazione seria, nella quale, poiché le regole vengono rispettate, si riesce anche a creare l'ambiente corretto per l'economia. Potrei fare molti altri esempi: strappare alla criminalità le zone franche, le periferie abbandonate o le Caivano di turno, come le tante altre periferie nelle quali, con l'operazione Alto impatto, il ministro Piantedosi, che voglio ringraziare, ed io ci siamo recati, vuol dire rimettere interi territori di questa Nazione a lavorare e a produrre nel rispetto delle regole. Significa rafforzare l'economia italiana e indebolire la mafia, la 'ndrangheta, la camorra e chi ha bivaccato su uno Stato che era debole.

non è una scatola chiusa, ma un disegno di legge a disposizione del Parlamento; sono certa e convinta che, grazie anche al lavoro che il Parlamento farà - e questo lo dico a tutte le forze politiche - il disegno di legge potrà essere rafforzato e diventare ancora più organico di com'è uscito dal Consiglio dei ministri.

questa questione legata al fatto che un'Italia più sicura significa anche un'Italia che vada nella direzione di una maggiore crescita economica è un tema che lei ha fatto molto bene a toccare, perché se ne parla poco, quindi è un elemento assolutamente importantissimo. Allo stesso modo, ci sentiamo di dire al Governo che bisogna anche avere pazienza, perché sappiamo che sulla questione c'è tanta aspettativa

alla fine ce ne saranno altri 1.400. Questo vuol dire che con tale approvazione l'anno prossimo si ripristinerà quel contingente che la sinistra aveva ridotto e diminuito con il Governo Conte-*bis*

il Gruppo Partito Democratico le pone quesiti sull'oggi, un oggi che incide pesantemente sul domani. Evitiamo di rifugiarci nel passato reciprocamente, provando a trovare alibi che oggi non servono a nessuno. Il disegno di legge di bilancio, signora Presidente, è iniquo e regressivo. Altro che fiducia a cui ha fatto riferimento prima: non c'è fiducia, signora Presidente, quando, mese dopo mese se lo faccia confermare dal ministro dell'economia Giorgetti - si emettono titoli di Stato con 50, 60, 70 *basis point* sulla Grecia e 100, 150 o 200 (purtroppo) *basis point* sugli altri grandi Paesi d'Europa. La La legge di bilancio prevede restrizioni sui requisiti e condizioni di accesso sui più deboli e soprattutto sulle misure di flessibilità in uscita come Ape sociale, Opzione donna e Quota 103.

Questa misura, in vigore dal 2017, è stata compressa escludendo dal diritto tutte le persone che sono nate dopo il 1o agosto 1951. È bene che chi ci ascolta a casa ne sia consapevole. Per Opzione donna, signora Presidente, nonostante i dibattiti e nonostante gli impegni assunti qui in Aula in queste ore, il requisito dell'età di accesso viene ulteriormente elevato. Signora Presidente, riguardo Quota 103 per il 2024 è previsto un abbattimento permanente della pensione. Si tagliano le pensioni. Non ci sarà una donna che accederà a Quota 103. *(Applausi)*. Vorremmo essere smentiti, signora Presidente, ma non ci sarà nel 2024 perché hanno hanno già perfezionato il requisito per accedere al pensionamento con Opzione donna nel 2021. Si realizza il paradosso che una misura annunciata come flessibilità in uscita per le donne finisce per discriminare proprio le donne. Le donne non sono protette, ma discriminate. La revisione determina anche tagli e riguarda 700.000 lavoratori pubblici. La retroattività non è costituzionale, signora Presidente del Consiglio.

del pensionamento, di fermarvi finché siete in tempo. Sopprimete l'articolo 33 del disegno di legge di bilancio che penalizza i medici italiani che

per la sopravvivenza dello stesso Servizio sanitario nazionale. Alla Presidente del Consiglio chiediamo che a questi lavoratori, ai 700.000 lavoratori e ai medici ogni giorno in trincea che combattono una battaglia per tutti noi, si dia oggi un segnale chiaro. Fermatevi e sopprimete l'articolo 33 del disegno di legge di bilancio. Signor Presidente, gli interroganti del PD chiedono ragguagli sulla tutela dei diritti acquisiti di chi è prossimo alla pensione. Io posso affermare che la legge di bilancio garantisce congruità sociale, equità dei regimi pensionistici, insieme chiaramente alla sostenibilità del sistema previdenziale. Voglio dire che noi abbiamo lavorato soprattutto per garantire in ambito pensionistico una tutela maggiore ai più giovani e a chi rientra interamente nel sistema contributivo. Per loro abbiamo eliminato l'ingiusto requisito, che fu introdotto dalla legge Fornero, per il quale chi era nel sistema contributivo aveva diritto alla propria pensione di vecchiaia solo quando questa era pari ad almeno l'1,5 per cento della pensione sociale; altrimenti, si sarebbe dovuto attendere addirittura fino ai 71 anni per poter maturare la propria pensione. Grazie a questo Governo, molti degli attuali lavoratori avranno diritto alla pensione a sessantasette anni, quindi quattro anni prima di quanto era previsto dal sistema attuale. Abbiamo confermato in gran parte le precedenti forme pensionistiche anticipate, che ricordo essere di natura sperimentale e che, diciamocelo anche qui, i precedenti Governi, compresi quelli dei quali facevano parte gli interroganti, non hanno mai inteso rendere strutturali. Però, a differenza di quanto fatto finora, noi non intendiamo proseguire nella prassi, un po' cinica, di aggravare oltre ogni limite di decenza la futura pensione di chi oggi è giovane. Questo perché io penso che un cittadino sia un cittadino indipendentemente dall'età che ha e che, come sempre, le tutele devono essere le più alte possibili, ma debbano essere uguali per tutti. A differenza di quanto fatto finora, noi sappiamo che questa Nazione ha bisogno, sul tema delle pensioni, di un intervento strutturale e non di misure estemporanee. Infatti, tra i nostri obiettivi c'è anche quello di procedere, nell'arco della legislatura, ad una riforma adeguata, strutturale, per dare ai cittadini le certezze dovute sul diritto di accesso alla pensione, secondo il principio di equità tra i lavoratori e tra le generazioni. Prorogando l'Ape sociale ed Opzione Donna, seppure con un aumento del requisito anagrafico, è stato confermato uno strumento di flessibilità in uscita, rispettando le esigenze, che ovviamente sono necessarie, di sostenibilità finanziaria di queste misure. La nuova quota 103 vuole ampliare le possibilità di pensionamento e favorire le soluzioni di uscita graduale dal lavoro. Per quello che riguarda l'articolo 33 della manovra, che coinvolge anche alcuni medici, come è stato chiarito in più sedi, si tratta di una misura che interviene su un particolare regime pensionistico di una parte di dipendenti pubblici, rispetto alla quale era stata evidenziata, da più parti, l'esistenza di un trattamento che era disomogeneo tra dipendenti e disomogeneo anche tra gli stessi medici. Su questa linea, del resto, si sono espressi anche economisti non sospettabili di essere dei sostenitori del Governo. In ogni caso, però, come lei saprà, il Governo ha già annunciato che intende rivedere la norma, con particolare riferimento proprio al tema degli operatori sanitari e che, in ogni caso, faremo in modo che non subisca alcun tipo di penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia e chi ha un'elevata anzianità contributiva.

presidente Meloni, non ci siamo. Anche sui medici, oggi era opportuno dire una parola chiara, perché ci sono migliaia di famiglie che, entro il 30 novembre, per vostra scelta, dovranno assumere una decisione. Andare o non andare in pensione? Questo sapendo che, se non vanno in pensione, perderanno una quota del loro trattamento pensionistico. Questo noi non abbiamo il diritto di negarlo, nessuno di noi. Presidente Meloni, il suo Governo sta tagliando le pensioni dei dipendenti pubblici, delle donne e dei medici costringendoli alla fuga. Se non arrivano parole chiare da questa giornata, sarà inevitabile la battaglia durante la legge di bilancio. State danzando, di promessa in promessa, non tanto sul Titanic, quanto sulle navi della Marina borbonica. Se le ricorda? Ogni giorno una *ammuina*, per far capire che ci siete; ogni giorno l'annuncio di un provvedimento che il giorno dopo verrà sconfessato. È più lungo l'elenco dei vostri dietrofront rispetto a ciò che il Governo ha fatto. Qualcuno di buon senso anche fra voi, Presidente vi dovrà informare che siete schiacciati dalle migliaia di ricorsi già partiti, perché i vostri pasticci sulle pensioni con i quali toccate diritti acquisiti, e malgrado i vostri sogni di premierato, inevitabilmente si schianteranno schianteranno contro una Costituzione solida. C'è ancora una Corte costituzionale nel pieno delle sue funzioni, signora Presidente e signor presidente La Russa, e sarà inevitabile, se calpestate la Costituzione, essere fermati inevitabilmente dalla stessa Carta costituzionale. Signor presidente La Russa, mi consenta solo un *tweet*, perché la Presidente del Consiglio ha parlato della piattaforma Sfinge. Quella piattaforma è stata modificata su richiesta del commissario Figliuolo - se lo faccia raccontare, signora Presidente *(Applausi)*- ed è stato fatto perché quella piattaforma, che ha funzionato consentendo cento per cento dei ristori del terremoto, è stata modificata perché avete scelto di nominare un commissario dopo tre mesi. Noi ci siamo e ci saremo sempre e comunque per tutti.

finestra") sul protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di immigrazione,

La riforma costituzionale, che abbiamo incardinato questa mattina, cambia quattro articoli della Costituzione, mentre in passato proprio il Partito Democratico ne aveva presentata una che ne cambiava quarantasei. Per cui direi che, se qualcuno deve avere prudenza, forse non siamo noi, ma sono altri. Venendo al tema, nel corso dei suoi tredici mesi di mandato come Presidente del Consiglio lei ha effettuato quarantotto viaggi internazionali ufficiali, stipulando accordi

in materia migratoria per contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori illegali e poter accogliere meglio gli aventi diritto alla protezione internazionale. È un testo che prevede, fra l'altro, che l'Albania fornisca gratuitamente all'Italia gli spazi per costruire dei centri per la gestione dei migranti in due località a 70 chilometri circa dalla capitale Tirana. Tra l'altro, quell'accordo è molto probabilmente sorto non in uno di quei quarantotto viaggi classificati come ufficiali, ma in quel viaggio, che alcuni hanno anche avuto il bel gusto di criticare, fatto a titolo privato nell'agosto scorso, visitando il primo ministro albanese Edi Rama. è la seguente: quali sono i vantaggi concreti per l'Italia derivanti da questo accordo e quali sono i riflessi rispetto all'Unione europea, che sono evidentemente anche da considerare?

e molto innovativo, che racconta uno spirito di cooperazione europea, e poi le dirò perché. È un accordo che nasce da alcune considerazioni condivise che io ho fatto con il primo ministro Rama - come lei ha detto correttamente - quando tutti quanti erano troppo impegnati a cercare di capire come avessi raggiunto l'Albania, per il ciclo "non ci hanno visto arrivare": tutti pensavano che stessi in vacanza e, invece, stavo cercando di arrivare a un obiettivo che per me era molto importante.

preziosa. Ho sentito - e mi dispiace - ogni genere di *fake news* su questo accordo. Ho compreso che vorremmo costruire una Guantanamo all'italiana, deportare i migranti, che l'accordo violerebbe il diritto internazionale. Ma vedete: l'unico diritto che l'accordo viola è quello dei trafficanti di esseri umani, che è stato garantito molto in passato, ma che certamente non garantirà questo Governo. Dopodiché, l'accordo rispetta ovviamente il diritto internazionale. I migranti non vengono deportati, perché banalmente l'Albania non è la Germania nazista, ma è un Paese, uno Stato di diritto candidato all'ingresso nell'Unione europea e presieduto, tra l'altro, da un *Premier* socialista; *Premier* che la sinistra italiana ha cercato di far espellere dal Partito socialista europeo perché evidentemente non è più di sinistra accogliere i migranti o forse banalmente non è di sinistra aiutare l'Italia. *(Applausi)*. Io penso che invece penso che invece il *premier* Rama abbia dato un grande segno di disponibilità. Semplicemente, quello che accade con questo accordo è che migranti soccorsi da navi delle autorità italiane possono essere condotti in centri gestiti in Albania con giurisdizione italiana; le procedure sono italiane, lì operano le nostre Forze dell'ordine, operano le nostre commissioni d'asilo. In quei centri si applica il diritto italiano, che è ovviamente anche diritto europeo. anche qui un'altra *fake news* che ho sentito dire, nel solito tentativo affannoso di cercare il soccorso esterno quando non si sa quali argomenti utilizzare in patria, è che l'accordo è in violazione del diritto europeo. Poi ha risposto direttamente l'Europa, con diversi interventi, l'ultimo dei quali è proprio quello del cancelliere Scholz di ieri, che l'accordo non viola le norme europee e anzi l'Europa è interessata ad approfondirlo. È ciò che accade sempre quando si fanno delle cose sensate. Si è detto anche che il Governo aveva esautorato il Parlamento. Non è nostra intenzione - il ministro Tajani, che ringrazio, lo ha già detto - esautorare il Parlamento, perché questo accordo chiaramente è una cornice. Ma noi sottoporremo in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche tutte le norme, quelle di spesa e di attuazione del protocollo. Anche il Parlamento, quindi, verrà coinvolto. Detto questo, voglio approfittare di questa occasione per ringraziare da quest'Aula il Primo Ministro albanese e l'Albania tutta per il grande aiuto che ha offerto all'Italia in un momento di difficoltà. *(Applausi)*. Credo che sia stato un atto di grande generosità e credo - permettetemi - che sia stata anche una grande lezione, soprattutto a chi ha sempre parlato di solidarietà europea senza di fatto mai riuscire a ottenerla. Oggi questo Governo ottiene solidarietà non solo dall'Europa, ma anche dai Paesi extraeuropei, perché fa proposte serie,

pienamente soddisfatto. Ci riteniamo pienamente soddisfatti soprattutto del lavoro fatto in questi tredici mesi, insieme a tutto il Governo, a tutti i Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari qui presenti, che saluto. Il nostro sostegno è naturalmente totale per l'impegno, la determinazione e le capacità che vediamo esplicare nell'azione di governo. In questi giorni qualcuno ha detto che Fratelli d'Italia ha un'impostazione patriarcale. Noi non sappiamo bene cosa si intenda, ma naturalmente le senatrici e i senatori di Fratelli d'Italia sono orgogliosi di sostenere la prima donna Presidente del Consiglio innanzitutto per la sua capacità, determinazione, impegno e abnegazione nel sostenere gli interessi degli italiani. Come definire questo non lo sappiamo: noi lo definiamo essere patrioti.

Presidente, ci ha donato la spilletta e a questo simbolo si aggiungono anche le scarpette rosse, il simbolo più importante della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza sulle donne. Per me era importante che questo simbolo trovasse spazio in quella che l'istituzione più rappresentativa della nostra Repubblica. Sono scarpette realizzate in ceramica a mano da una ceramista del mio paese. Speriamo che questi simboli incentivino le donne a chiedere aiuto e a denunciare. La ringrazio, Senatrice, io la ringrazio e con lei ringrazio la vice presidente Castellone, che è la vera ideatrice dell'occasione di ricordare in maniera commossa le tante, troppe donne cadute innocenti sotto la violenza degli uomini.